dirò resti a verbale dei nostri lavori come forma d'interpretazione autentica.

definiscono, secondo le norme dei loro Statuti, le città e le aree metropolitane e determinano il conseguente comportamento per la creazione delle stesse. Presidente, concordo con la precisazione quanto mai opportuna del presidente Vizzini. Ovviamente le Regioni a Statuto speciale provvedono, in questa materia, nei limiti della loro competenza e quindi, poiché si tratta, nella fattispecie, di norme di indirizzo, è chiaro che c'è un obbligo delle Regioni a conformare, nell'ambito delle loro competenze,

Ribadisco una posizione generale, che ho più volte espresso, ovvero che sarebbe stato necessario dedicare alla Carta delle autonomie un impegno prioritario, e quindi sciogliere qui tutti i nodi, compreso quello della città metropolitana. Abbiamo invece intrapreso un'altra strada, che è stata quella d'inserire comunque in questo testo alcuni aspetti anche attinenti alle funzioni di Comuni e Province ed alla attribuzione di competenze,

relativo ai finanziamenti) che quindi può essere incentivato, noi abbiamo alla fine convenuto su questa posizione. Questo testo, peraltro, può rappresentare un elemento di opportunità: tutti sappiamo che da decenni si discute delle Città metropolitane, che sono previste nella nostra Costituzione, e mai si è addivenuti ad una loro istituzione. Vi è una normativa vigente, che peraltro non ha mai trovato attuazione, la quale parte dal fatto che occorre un'intesa tra Comune capoluogo e Provincia per dare avvio alla procedura istitutiva della città metropolitana.

E allora, abbiamo proposto tre ipotesi di avvio: da un lato, quella dell'intesa, così com'è a legislazione vigente; dall'altro, quella della promozione del Comune capoluogo,

contemperata dallo stesso peso dei Comuni, sia numerico, sia relativo alla popolazione. Credo quindi che si sia data un'opportunità, anche con una certa competitività, per avviare questo processo, che però riteniamo debba essere condotto con grande democrazia, tant'è vero che l'ipotesi referendaria consentirà ai cittadini tutti di esprimersi sulla procedura. Voglio chiarire che il nostro voto favorevole attiene ad un processo di carattere provvisorio: non andiamo qui a normare la città metropolitana e siamo molto impegnati - questo hanno dichiarato il ministro Maroni e il sottosegretario Davico - a trovare una soluzione nella Carta delle autonomie

Ci sembrava molto squilibrato e poco sostenibile il fatto che queste opportunità non fossero parimenti garantite alle altre realtà che, a normativa vigente, possono costituirsi in Città metropolitane, per quanto riguarda

le funzioni definitive, cioè fondamentali delle Città metropolitane, perché, così come abbiamo detto per i Comuni e per le Province, altrettanto coerentemente dobbiamo fare per le Città metropolitane. quindi, una prima individuazione delle funzioni di carattere provvisorio, che servono per la definizione dei finanziamenti

ha la sua normativa, altrettanto provvisoria e transitoria, nell'articolo a lei dedicato. Questo, quindi, è assolutamente importante, proprio per quella necessità di equilibrio e pari opportunità istituzionale alla quale mi sono richiamata. Tutta questa normativa dovrà trovare il superamento nella normativa di carattere definitivo. Credo che questo chiarimento, che è la motivazione vera della mia dichiarazione di voto positiva per il Gruppo del Partito Democratico, fosse dovuto perché è evidentemente un processo legislativo, da un lato, di grande complessità e, dall'altro, oserei dire, di grande determinazione nel raggiungere determinati risultati di futuro istituzionale, ma anche di concretezza prendendo atto del quadro istituzionale attuale.

su questo articolo aggiuntivo. Cercherò di tenermi basso: l'argomento si presta a moltissime osservazioni anche teoriche che risparmierò. Le perplessità vertono intanto su una questione di metodo che, sia pur brevemente, non posso fare a meno di accennare e cioè che, dopo mesi di discussione molto articolata e molto interessante su tutto il provvedimento, se questa era una lacuna (e in un certo senso lo era), ce ne si poteva rendere conto prima e si poteva cercare di discutere con meno precipitazione. Adesso ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo discutere sotto il pungolo del tempo che fugge questo nuoce anche alla chiarezza degli elementi in discussione. Mi limito ad osservare che, benché inserito in Costituzione, il termine «Città metropolitane» è ben lontano dall'essere stato chiarito nella sua natura. L'osservazione fondamentale è che, mentre le istituzioni le istituzioni esistenti (Regione, Provincia, Comune), al di là della loro natura concreta, hanno anche un certo carattere astratto, nel senso che sono istituzioni della comunità civile quindi, esistono indipendentemente dai loro confini (ne hanno, ma la loro natura intima di istituzioni della società civile prescinde dalla fisicità del luogo), la città metropolitana è una sorta di ibrido tra un'istituzione e un'entità concreta; la città metropolitana è un insieme urbanistico

Questo già pone un problema difficilissimo di individuazione dei soggetti. Si potrebbe chiedere (credo con estrema facilità), sentendo uno o due urbanisti di opinioni diverse,

meno, senza nuocere a nessuno, perché la città metropolitana deve essere qualcosa di molto vasto, ramificato, esteso in uno spazio apprezzabile e che ponga dei problemi di coordinamento non solo territoriale, ma anche socio-economico. quindi, l'oggetto stesso che sfugge; non c'è nemmeno una bibliografia sufficiente per affrontare questo tema e rischiamo di dare una definizione provvisoria di una cosa che invece, per essere definita e individuata, avrebbe bisogno di molta più dottrina, di molta più analisi e di un esame molto più ravvicinato. Si rischia poi, nell'esame degli elementi particolari, di rilevare delle stranezze. esempio, nel caso in cui la Provincia venga sostituita da una città metropolitana, non si capisce bene quali siano le garanzie che determinano un mutamento in positivo. Provincia era, città metropolitana diventa; gli organi decadono e vengono cancellati però sostanzialmente, ad uno sguardo disincantato, ciò appare come una sorta di sostituzione: organi che erano della Provincia diventano organi della città metropolitana, ma non se ne coglie la ragione progressiva. Un elemento di confusione nasce dal fatto che che possono essere previste Città metropolitane costituite dalla non totalità dei Comuni della Provincia che rinuncia a sé stessa, dunque bisogna immaginare che i Comuni passino ad altre Province. La questione dei limiti delle spese, poi, è ambigua, perché, mentre da un certo punto di vista sembra di poter capire che l'obiettivo è quello di non aumentare i costi, al comma 7 dell'emendamento 21.0.100 (testo 2) si dice invece che il finanziamento «assicura loro una più ampia autonomia di entrata». cosa vuol dire autonomia di entrata? Più soldi o, invece, più autodeterminazione nel gestire i soldi che ci sono? Insomma, mi rendo conto che affastello con difficoltà - perché questo argomento necessiterebbe di essere affrontato con maggiore cognizione di causa - elementi eterogenei,

questa è una buona intenzione, se si riesce a darle effetto, o perlomeno è una garanzia di non aggravio sistematico e crescente. Un'ulteriore garanzia la si può trovare, come l'ha trovata la collega Bastico,

luci ed ombre ed io non volevo tacere le ombre perché fanno parte di un quadro effettivamente piuttosto opaco su cui contiamo, attraverso uno sforzo

Signora Presidente, esprimo parere contrario

Stiamo votando la riforma dell'ordinamento della capitale in un disegno di legge sul federalismo fiscale. fiscale. Ci troviamo di fronte alla conclusione, a suo modo razionale, di un processo politico che vede, cari nell'approvazione di questo disegno di legge molte convenienze, definire un compromesso di sistema, ma anche non risolvere una serie di problemi che poi saranno sottolineati nella Il tema della capitale però è rilevantissimo. L'articolo 114 della Costituzione recita: «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento». Questa è la legge dello Stato che disciplina l'ordinamento della capitale: molti colleghi non se ne sono resi conto. Sottolineo che, tra le cose rilevanti che avvengono con questa votazione che stiamo per assumere, vi è la soppressione del Comune di Roma, la soppressione del Consiglio comunale di Roma. Ciascuno di noi in quest'Aula potrebbe ripercorrere vicende storiche (non lo faccio nei brevissimi minuti che ho a disposizione), ma non vi sfugge che

subentra attraverso una normativa che non ha la dignità di essere approvata dal Parlamento della Repubblica. si occupa della capitale della Repubblica e legifera sull'ordinamento della capitale della Repubblica come stabilisce la Costituzione, ma, come sintesi di un compromesso che ha riguardato le isole,

dell'ordinamento della capitale nel disegno di legge sul federalismo fiscale. Lo facciamo con una manovra che non è «malaccio» - lo dico esplicitamente - e contiene alcune parti positive, ma segnalo ai colleghi che, a sostegno della richiesta di stralcio avanzata dal Gruppo dell'IdV che sarà sostenuta dal Gruppo del Partito Democratico, questo compromesso tra le convenienze si configura, signora

all'Assemblea, ci troviamo con una definizione che non è propria di un testo di legge e tanto meno di un testo di legge di rango adeguato al recepimento di una norma costituzionale. Tra

L'intervento dei nostri colleghi, anche su sollecitazione di alcuni di noi, ha fatto sì che si modificasse la norma ancora più assurda che era stata definita si riferiva alla tutela del patrimonio culturale-storico-artistico. Considerate che è materia indisponibile per gli enti locali, come lo è per le Regioni, perché è assegnata allo Stato; anche la definizione, colleghi, di valorizzazione di beni storici, artistici ed ambientali. Una norma di quel tipo che avrebbe stabilito che l'ente locale avrebbe nella capitale la competenza, solo per fare un esempio, della valorizzazione del Quirinale.

condividiamo buona parte dei temi di merito che, anche grazie alla nostra battaglia, sono stati sensibilmente modificati, anche rispetto alle incomprimibili potestà legislative della Regione Lazio ed alla prospettiva testé illustrata della città metropolitana. Riteniamo che il modo più razionale per affrontare questa materia, che è bene il Senato affronti - e come vediamo i tempi sono abbastanza maturi - sia quello di approvare oggi il disegno di legge sul federalismo fiscale, ma di approvare mi viene da dire - come Parlamento comanda, le norme sulla capitale della Repubblica in uno specifico provvedimento che si adotti da parte della Camera e del Senato con la giusta attenzione, meditazione e - permettetemi - con una qualità adeguata alle norme di cui stiamo discutendo. *(Applausi

che riguardano la determinazione del territorio e dei confini della città ed il rapporto tra la città ed il territorio della sua Provincia perché è in questa veste che si deve non può affrontare, ad esempio, il tema che può essere oggetto di una norma costituzionale - su questo abbiamo presentato una proposta di legge - che riguarda anche il sistema istituzionale di Governo e l'autonomia normativa che la capitale del nostro Paese deve avere per garantire la qualità del Governo del suo territorio e dell'interesse anche internazionale che su questo territorio c'è. Questi temi non possono essere affrontati un quarto d'ora prima della votazione finale di questo provvedimento e solo perché magari serve a qualcuno fare qualche conferenza-stampa fuori da questo Palazzo per dire che il federalismo fiscale si è occupato anche di Roma capitale. Roma è un tema troppo serio per essere affrontato in termini così ridotti, minimalisti e - se mi consentite - inutili se non ad alimentare una propaganda che penso sia finita da tempo e che ci dovrebbe tutti portare invece a confrontarci in Parlamento su come migliorare il sistema di Governo

l'intervento. Anche quel caso è la testimonianza vivente di una non scelta, cioè della scelta di non decidere cosa fare delle Province e delle aree metropolitane, che nei territori interessati sono sovrapposte. La scelta di non scegliere significa sostanzialmente produrre un ulteriore risultato negativo,

fin qui fatto in relazione ad un avvenimento che definisco storico. Finalmente questo Parlamento, senatore Rutelli, si occupa della sua capitale e lo fa con un provvedimento che è all'attenzione di tutto il Paese, un provvedimento nel quale sicuramente questa vicenda di Roma capitale ci sta e ci sta anche per segnare una sua differenziazione. Sento ripetutamente alcuni colleghi che si riferiscono alle Città metropolitane e c'è un articolo 21 che poco fa abbiamo approvato in relazione a tale vicenda,

è una fattispecie che finalmente identifica la capitale; accadde sette anni fa e noi soltanto oggi, a sette anni distanza, legiferiamo in relazione a quel comma dell'articolo 114 e lo facciamo giustamente e con proprietà. Potremmo fare di più e meglio; non ho dubbi che si potrà fare di più, ma a partire da questo gesto verso la capitale che - ricordo - è la città più grande d'Europa, ma non per dire che è l'uomo più alto del mondo, ma esattamente il contrario. Qui siamo di fronte

che questa città capitale non ha una *governance* adeguata dal 1948. Oggi, oltre a tutto il resto, noi diamo una *governance* alla capitale d'Italia, grazie a questo Parlamento ed a questo Governo, che ha ritenuto di volerlo fare velocemente proprio in questo provvedimento che riguarda anche il federalismo del nostro Paese. Per tale ragione, penso che stiamo facendo qualcosa di importante. importante. Anche i sindaci che hanno preceduto la giunta Alemanno hanno tentato di fare qualcosa del genere, soprattutto il sindaco Veltroni. Il Governo Prodi non riuscì a dare attuazione alle richieste di Campidoglio del suo sindaco. Oggi questo Governo lo fa. Grazie di nuovo.

contenuto nella delega al Governo sul federalismo, anche perché in tal modo l'articolo risulta estraneo per materia al federalismo fiscale e generico nella sua formulazione. Riteniamo maggiormente proficuo rimandare l'intervento normativo ad una disciplina specifica ed autonoma la quale possa, a seguito di una più approfondita riflessione, strutturare in materia organica e completa l'architettura economica ed istituzionale di Roma capitale. Se l'ordinamento di Roma, infatti, fosse caratterizzato da genericità e confusione, come avverrà sicuramente tramite l'inserimento dello stesso nella legge sul federalismo, si potrebbero creare dinamiche poco virtuose, lo spreco di risorse, lo stallo gestionale o ancora l'irresponsabilità politica della classe dirigente. È giusto delegare poteri a Roma e al suo territorio limitrofo, in quanto solo se le decisioni partono da istituzioni più vicine ai cittadini diviene possibile governare in maniera più efficiente a livello economico e più efficace a livello politico. Questo è il principio della sussidiarietà, che anche l'Europa promuove, ma la questione è quanto bisogna delegare e come. I punti focali dell'ordinamento di Roma capitale devono sciogliere diversi interrogativi

però, si legge al comma 9 che, a decorrere della istituzione della Città metropolitana, le disposizioni dell'articolo si intenderanno riferite alla Città metropolitana di Roma. Quindi, a nostro avviso, è errata la riflessione del senatore Cutrufo, che è poi anche vice sindaco

il senatore Rutelli. Esse vogliono semplificare e fondono gli uffici comunali con quelli provinciali ed assorbono gli interessi di natura sovracomunale in quanto hanno competenze sul comune di Roma e su quelli limitrofi. Di conseguenza, potrebbe scaturire una possibile confliggenza dalla configurazione dell'ordinamento di Roma capitale, così come nella delega, a quella a seguito della introduzione della Città metropolitana con conseguenze negative nella gestione dei servizi essenziali. ad esempio ai trasporti: sarà una conduzione integrata dell'area o la gestione sarà divisa fra Comune, area metropolitana, Provincia? In secondo luogo, si deve considerare la questione finanziaria. Nel testo si legge che alla città di Roma verrà attribuito un patrimonio proprio commisurato sulle funzioni e competenze ad essa attribuite e derivante, fra le altre fonti, dal trasferimento, a titolo gratuito, a titolo gratuito, dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale. Tuttavia, una simile disposizione, senza la specifica di criteri aggiuntivi, rischia di portare ad una cartolarizzazione fatta alla buona. fatta alla buona. Si rischia di regalare al Comune beni dello Stato senza specificare quali beni gli si vuole concedere (il Colosseo, per esempio, paradossalmente), senza specificare chi decide, senza indicare i principi di scelta. onorevoli colleghi, a quanti abusi e a quante malversazioni possono essere fatte nel dismettere beni statali senza un controllo puntuale! Sempre a livello finanziario, se le disposizioni contenute in questo provvedimento si leggono in combinato con quanto affermato dall'articolo 18, comma del cosiddetto decreto salvacrisi (Atto Senato n. 1315) dove si stabilisce che il Comune di Roma è escluso dall'applicazione del Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010, allora la possibilità che lo scopo del federalismo (ossia l'efficienza economico-amministrativa, come recita il ministro Calderoli) venga totalmente vanificato, nel caso di Roma diventa tangibile! Il terzo ed ultimo punto riguarda l'attribuzione delle funzioni amministrative a Roma capitale. Anche la suddivisione delle competenze non è scevra da controversie in quanto si deve mantenere l'equilibrio fra la puntuale definizione delle stesse per evitare vuoti decisionali e la necessaria elasticità che deve mantenersi per permettere una modifica allorquando sorgano nuove necessità che possano essere affrontate meglio a livello locale piuttosto che nazionale. Allora, cari colleghi, è opinione dell'Italia dei Valori che sia necessario stralciare stralciare dalla legge delega la disposizione che disciplina l'ordinamento di Roma capitale e di trasferire il provvedimento ad un testo specificatamente dedicato a ciò,

Colleghi, restate seduti. Relatore Azzollini, le do il tempo perché lei possa prendere la tessera.

compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Pertanto, questo rischio non c'è, è il combinato disposto che lo elimina.

alcune piccole modifiche del testo, la più rilevante delle quali, che attiene ai pareri della Commissione bilancio, è stata ampiamente illustrata a tutta l'Assemblea, che ne è a conoscenza. Pertanto, il parere del

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi del Senato della Repubblica, il Movimento per l'Autonomia, sin dall'avvio del dibattito politico sul tema del federalismo e su questa importante riforma, ha assunto un atteggiamento di grande apertura, senza farsi trascinare in atteggiamenti di impaurita autoconservazione, superando analisi banali che considerano questa, che noi valutiamo un'opportunità, un pericolo per l'unità del Paese. Paese. Lo abbiamo fatto per due ragioni distinte. La prima è nella stessa ragione fondativa del nostro movimento, *nomen omen*. Un movimento che pone a suo fondamento il valore dell'autonomia dei territori e della loro responsabilità di autogoverno non può che guardare con fiducia ad una riorganizzazione dello Stato che metta al centro

su quello che è il precipitato di 150 anni di falsa unità nazionale e di mancata applicazione dei princìpi della Costituzione repubblicana. Qualsiasi indagine o rigorosa analisi scientifica conferma ogni giorno che questo è un Paese spaccato, drammaticamente lacerato, in tutti gli indicatori, sia che essi guardino al reddito *pro capite*, alla dotazione infrastrutturale, alla qualità dei servizi o al numero delle imprese che agiscono nel territorio. Di cosa dovremmo aver paura noi del Mezzogiorno? Di quello che viviamo ogni giorno, della nostra drammatica realtà? dicevo, è il frutto di una falsa unità nazionale, oltre che di una mancata applicazione dei princìpi della Costituzione, di cui sono parte integrante gli statuti autonomistici delle Regioni a Statuto speciale, concessi da uno Stato formalmente generoso, che li ha però svuotati, contrastandoli con la sua impostazione centralista e confidando anche nell'ignavia e nell'incapacità delle classi dirigenti locali, che non hanno mai assunto il valore dell'autonomia come riferimento reale della loro azione politica. Il nostro movimento nasce per questo: nasce per colmare questa lacuna storica e politica e per assumere il valore della responsabilità dei territori come principio essenziale dell'azione politica; per contrastare - una politica centralista che ha scelto di rimuovere il tema del Mezzogiorno e del suo ritardo di sviluppo

qualche protagonista di quella stagione politica siede in questo Parlamento - in cui la politica nazionale assunse un'iniziativa per fronteggiare questa drammatica emergenza economica e sociale, attraverso l'intervento straordinario. L'intuizione era apprezzabile; la prassi operativa fu un fallimento, un disastro. Era un'operazione centralista che produsse sprechi, inefficienze ed anche malaffare. Ma ad una politica fallimentare si è sostituita l'assenza di qualsiasi politica. Oggi, di fronte ai nostri concittadini, noi vogliamo assumere in pieno e direttamente la responsabilità delle politiche del nostro sviluppo. Per questo stiamo compiendo scelte coraggiose, improntate al rigore, all'efficienza ed alla trasparenza. Vogliamo togliervi

giudizi che consentono ai ceti dirigenti di questo Paese, spesso assistiti ben più del Sud, di marginalizzare il problema, di rimuoverlo, concedendoci qualche intervento di politica assistenziale che viene accompagnato da un disprezzo intellettuale. Non abbiamo bisogno di questo. Per questo noi faremo la nostra parte, ma pretendiamo rispetto, pretendiamo i nostri diritti, pretendiamo il giusto. Il federalismo dovrà essere equo e solidale e la perequazione dovrà costituire un obiettivo reale e prioritario, a cominciare da quella infrastrutturale, per continuare con la possibilità di una fiscalità differenziata, sino ad una rinegoziazione delle entrate, prime fra tutte quelle derivanti dalle accise sugli idrocarburi raffinati nei territori regionali. I princìpi di queste scelte sono tutti contenuti nella legge delega, ma si tratta di princìpi - perché questa è una legge delega - che vanno riempiti di contenuti.

assegnamento sulle energie del territorio e noi questa sfida la raccogliamo, confidando nel valore delle nostre comunità e anche - vi confesso - nella voglia di riscatto di queste comunità. Se deve esservi, attraverso il federalismo, una competizione virtuosa dei territori sul terreno dell'efficienza, tutti debbono essere messi nelle condizioni di un confronto aperto. Noi del Movimento per l'Autonomia sappiamo di poter contare su un Governo che già nella fase di elaborazione di questo progetto di legge delega in Commissione si è reso disponibile ad un confronto costruttivo, con la flessibilità di chi vuole riformare lo Stato, ma sa di non poterlo fare in solitudine: di offrirsi ad un confronto impegnativo, in cui tutti i contributi hanno pari dignità, certamente rispettando l'intuizione e la vocazione politica del Governo. In questo riconosco all'Esecutivo, ed in modo particolare agli uomini della Lega, il merito di avere imposto questo tema nell'agenda di Governo, anche perché sollecitato dalle tensioni, dalle motivazioni di aree molto forti del Paese, insoddisfatte di quella che oggi è la capacità del Governo centrale e della sua burocrazia.

dello Stato, assumendo questa responsabilità di fronte alla nostra gente, che speriamo si apra con fiducia rispetto alla nostra azione politica e che superi anche lo stretto confine del Mezzogiorno, perché quello dell'autonomia è un valore che

Il nostro vostro favorevole, amici del Governo, alla legge delega sul federalismo fiscale non è una delega in bianco, ma un impegno reciproco ad un lavoro comune per scrivere insieme il nuovo patto civile e politico della nostra comunità nazionale e realizzare finalmente una vera unità del Paese.

Falso, perché così com'è non serve a contenere e a razionalizzare la spesa pubblica; non sappiamo infatti chi fa che cosa, perché non avete voluto definire chiaramente i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini italiani, né le funzioni fondamentali degli enti locali. Non sappiamo poi quali sono le altre funzioni che, in base alla Costituzione, devono essere attribuite a Regioni ed enti locali, perché non avete voluto scriverle nel provvedimento. Non lo avete fatto, perché avreste dovuto dire subito agli italiani quanto costerà caro il vostro federalismo fiscale. Il ministro Tremonti, ieri, in quest'Aula, ha detto che quello che avete creato è un sistema complesso con un numero elevatissimo di variabili: 12 tributi in gioco; 5 soggetti istituzionali che decidono; 11 criteri direttivi; 2 fondi statali; 8 procedure attuative. Questi sono gli unici numeri che il ministro Tremonti ha dato. Iniziamo ad interrogarci se in futuro, con questo federalismo fiscale, saranno ancora utili un Ministro per l'economia ed una legge finanziaria che non ha più ragione di esistere. Uncongegno ad alta complessità istituzionale, lo ha definito il ministro Tremonti, del quale è difficile valutare l'impatto economico. Secondo voi, quindi, i conti devono essere fatti dopo e non prima di affidare a Regioni ed enti locali così ampi poteri di spendere e di tassare. Secondo noi è pura follia. Ciò che chiedete al Parlamento è una vera e propria delega in bianco e ciò che chiedete al Paese è un vero e proprio salto nel buio. Eppure, l'articolo 119 della Costituzione, cui volete dare attuazione, vi obbliga a garantire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche delle Regioni e degli enti locali, senza il quale non vi è federalismo fiscale perché non vi è certezza dell'autonomia di entrata e dell'autonomia di spesa. Su questo provvedimento vi sono quindi tanti dubbi e pochissime certezze, e queste tutte in negativo. È noto che l'Italia ha un debito pubblico tra i più elevati al mondo ed è quindi costretta a pagare consistenti interessi. A questi deve far fronte lo Stato, sempre e comunque, pena l'inaffidabilità internazionale del Paese e le inevitabili ricadute negative per i risparmiatori che investono sul nostro sistema economico e finanziario. Chi si fa carico del debito pubblico? Nel provvedimento non ne parlate. A voler essere ottimisti è facile prevedere che lo Stato, oltre a finanziare le sue funzioni, dovrà giustamente onorare il pagamento degli interessi sul debito e quindi non potrà ridurre la pressione fiscale. Per garantire l'equilibrio dei conti pubblici tenterà poi di spogliarsi di quante più funzioni possibile, trasferendole a Regioni ed autonomie locali. Le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, a loro volta, non potranno ulteriormente indebitarsi - cosa buona e giusta e quindi saranno costretti ad aumentare le tasse per coprire vecchie e nuove funzioni. Altro che semplificazione e riduzione della spesa pubblica! Altro che equilibrio dei conti pubblici! Siamo al rischio dell'anarchia fiscale. In compenso avete moltiplicato i centri di spesa sovrapponendo alle Province le aree metropolitane, anch'esse con il potere di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. E come è finita con la soppressione delle Province? Era un vostro cavallo di battaglia in campagna elettorale. Altro che sopprimerle! Anche a loro più potere di tassare e di spendere. Avete già dimenticato i guasti che la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione ha prodotto nel rapporto tra Stato e Regioni e la crescita eccessiva di tutti i livelli territoriali della pubblica amministrazione, ivi comprese le cosiddette caste nazionali, regionali e provinciali. Questo è un federalismo fiscale falso, perché anziché ridurre la spesa pubblica e la pressione fiscale aumenta gli enti che spendono e tassano indiscriminatamente. Ed il sistema, quindi, per stare in equilibrio dovrà aumentare la pressione fiscale. Vi avevamo proposto un emendamento al riguardo, uno dei tanti che ci avete bocciato, che anche il senatore Baldassarri, presidente della Commissione finanze, ha votato con noi. Il vostro no è stato più eloquente del silenzio del ministro Tremonti sui conti pubblici. Noi abbiamo un'idea diversa del federalismo fiscale e del rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali e ve l'abbiamo proposta con i nostri emendamenti, contro cui avete votato: competenze e funzioni chiare e nette dello Stato, delle Regioni e delle autonomie; corrispondenza tra autonomia e decentramento delle funzioni amministrative, da un lato, ed autonomia di entrata e di spesa, dall'altro; ruolo insostituibile dello Stato nella perequazione e nelle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale; una proposta né populista, né disgregatrice dell'unità giuridica ed economica della Nazione, così come vuole la nostra Costituzione. Il vostro è anche un federalismo fiscale pericoloso. Il primo pericolo è il modo in cui avete cercato di definire il costo standard. Per carità, il superamento della spesa storica come elemento che regola i rapporti finanziari dello Stato con gli enti territoriali è condivisibile, ma il costo standard deve essere depurato delle inefficienze della pubblica amministrazione e tenere conto delle differenze territoriali, economiche ed infrastrutturali che incidono obiettivamente sui costi sopportati dalle imprese e dalla pubblica amministrazione. La differenza tra costo standard e costo reale, cioè il costo che sostengono le imprese e le pubbliche amministrazioni in diverse aree del Paese, lo caricate sui cittadini che, a prescindere dal reddito, saranno costretti a pagare più tasse perché vivono in parti svantaggiate del Paese. un federalismo iniquo, che divide il Paese perché gli strumenti che garantiscono il riequilibrio economico e sociale tra Nord e Sud sono a copertura incerta, sfuggono alla decisione e al controllo dello Stato e del Parlamento, come previsto dalla Costituzione e sono affidati alle decisioni delle Regioni più forti. Inoltre, con il provvedimento in esame scardinate tutti i sistemi di programmazione economica affidando a quattro Ministri (casualmente tre del Nord) il potere di decidere dove si fanno le infrastrutture e con quali risorse. Avete avuto anche il coraggio di chiamare questa operazione di potere in danno del Mezzogiorno perequazione infrastrutturale! L'unico esempio vivente di federalismo istituzionale e fiscale è quello che regola il rapporto tra Stato e Regioni a Statuto speciale. Avete demolito anche questo stabilendo che lo Stato decide unilateralmente le questioni finanziarie fondamentali per i bilanci delle Regioni autonome. Un federalismo fiscale debole con i forti e forte con i deboli, che non vi fa onore e che non serve al Paese. Serve solo alla Lega, che dopo il fallimento della secessione del 1996, della devoluzione del 2001 e delle Regioni a due velocità nel 2006 ha bisogno di dire qualcosa di federalista ai suoi elettori. La delega in bianco chiesta dal Governo serve solo a questo. C'è chi ha deciso di fidarsi di voi, sbagliando. Noi dell'UDC, no, e votiamo contro, nell'interesse del Paese.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il nostro Paese avverte l'esigenza indifferibile di essere più moderno ed agile, non solo nelle istituzioni, ma soprattutto nel modo di rispondere positivamente e tempestivamente alle istanze dei cittadini. Riforme, quindi, non da fare in riunioni al caminetto o attraverso la stampa o con una convegnistica spesso autoreferenziale; riforme in Parlamento, che che è il luogo per discutere, approfondire, contestare, contrastare, trovare soluzioni condivise. Certo, in molti ci rimproverano perché ci sono altri problemi, altre priorità, ossia le difficoltà delle famiglie, l'occupazione in decremento, le imprese in difficoltà. Su questi temi l'Italia dei Valori incalzerà il Governo senza nessuno sconto, ma dobbiamo lavorare - e le Camere devono farlo - su un piano interdipendente. Proprio in questa fase di crisi profonda, che certamente - ce lo auguriamo tutti - troverà un punto conclusivo, il nostro Stato alla fine deve trovarsi pronto a ripartire praticando il cambiamento virtuoso e superando una vecchia prassi. Ed è in un periodo di difficoltà che è giusto mettere a fuoco il festival degli sprechi a cui, soprattutto a livello territoriale, abbiamo assistito: ospedali costruiti, ma non consegnati e non funzionanti; strade ultimate, ma non collaudate; opere pubbliche senza manutenzione perché nessuno ne riconosce la proprietà; società a capitale pubblico fuori mercato, che erogano servizi a tariffe esorbitanti per il cittadino; costi della politica fastidiosi, al limite della insopportabilità per chi fatica ad arrivare alla fine del mese. Queste sono alcune delle motivazioni che hanno indotto l'Italia dei Valori come partito e il nostro Gruppo al Senato

dando il nostro contributo al miglioramento del testo senza rinunciare a vigilare sulla garanzia dei valori costituzionali quali l'autonomia, la solidarietà, l'efficienza, la responsabilità e la trasparenza. Ci siamo mossi - a tale proposito ringrazio con orgoglio i colleghi del Gruppo per il lavoro svolto - nella piena consapevolezza di voler dare attuazione alla riforma costituzionale del 2001 e della grande opportunità, attraverso il passaggio dalla spesa storica ai costi standard, e dunque alla valorizzazione del binomio autonomia‑responsabilità, per mettere in moto un processo positivo che porti maggiore efficacia ed efficienza all'amministrazione pubblica nel suo complesso. nel suo complesso. Peraltro, in presenza di un quadro istituzionale indefinito con riguardo alla distribuzione delle funzioni tra i livelli di governo e, soprattutto, con le grandezze finanziarie, i numeri e i costi di questa riforma non quantificati, né quantificabili secondo il Ministro dell'economia

con cui si dividono e si intrecciano le decisioni tra la capitale politica e i centri territoriali, i rapporti tra le Regioni e le comunità locali minori, la disponibilità delle risorse finanziarie per i servizi pubblici e, in fine e in principio, la garanzia di uguali diritti civili e sociali per i cittadini. la vita quotidiana degli italiani non cambia molto se il sistema elettorale maggioritario proporzionale è alla tedesca o alla spagnola, oppure se si forma un partito di centrosinistra con le primarie o una confederazione di centrodestra per volontà sovrana. La quotidianità dei cittadini risente moltissimo del livello di efficienza dei servizi pubblici, dunque

Il rispetto dei princìpi costituzionali non deve essere soltanto declinato. Noi riteniamo che la delega che parte da questo ramo del Parlamento sia ancora troppo generica, per cui bisogna verificare ancora i punti di dissonanza tra il disegno di legge in esame e la logica intera della nostra Carta costituzionale. Occorre poi accompagnare, o meglio inquadrare, il provvedimento con altri urgenti processi di riforma, come il superamento dell'attuale bicameralismo attraverso la creazione di una Camera delle autonomie territoriali o Senato delle autonomie, o come la chiameremo.

con la nuova Carta delle autonomie e con l'abolizione delle Province, che riteniamo essere un punto fondamentale. Rimangono ancora indeterminate la quantificazione e l'individuazione dei costi standard. Siamo certamente a favore del superamento della spesa storica, ma abbiamo necessità di capire se ciò avverrà in misura uguale in tutto il territorio nazionale, al netto quindi delle inefficienze e degli oneri aggiuntivi che possono manifestarsi in un determinato contesto territoriale. il vero nodo politico risiede nella determinazione dei costi standard. Nel testo non si rinvengono a questo proposito modalità e criteri puntualmente definiti. è poi quella che dichiaro essere la reticenza dei numeri, ministro Calderoli, a cui va il ringraziamento del nostro Gruppo per la disponibilità che ha manifestato in questi mesi. Il progetto del federalismo fiscale ha però, per sua natura, un profilo di ordine matematico, con ricadute di natura economico-finanziaria, perché le formule giuridiche rimandano a calcoli e numeri che vogliamo conoscere. Il Parlamento non può rimanerne all'oscuro. Le nostre proposte all'oscuro. Le nostre proposte emendative si sono mosse intorno ad alcune linee fondamentali: il rafforzamento del criterio di responsabilità la valorizzazione del principio di solidarietà in connessione con quello dell'unità nazionale. A tale scopo abbiamo voluto riconoscere il contributo fornito dalle diverse realtà locali alla creazione di ricchezza nazionale. Questo era il contenuto di un nostro emendamento che non è stato accolto e su cui invitiamo il Governo a riflettere, introducendo forme di indennizzo per situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione da parte di singole realtà territoriali di oneri e impegni nell'interesse di tutta la collettività nazionale.

corretta la perdurante fumosità rispetto ai princìpi e ai criteri direttivi, ai tempi, al quadro istituzionale di riferimento e, soprattutto, alle incertezze delle grandezze finanziarie. dell'Italia dei Valori ha deciso di esprimere un voto di astensione che si sostanzia in un segnale di fiducia nei confronti del e, allo stesso tempo, di monito, stimolo e controllo e - se me lo consentite, colleghi - di sensibilità istituzionale verso una riforma cardine per l'ordinamento italiano. Ma sfidiamo il Governo a migliorare la riforma nell'altro ramo del Parlamento. Saremo certamente sentinelle attente per impedirne degenerazioni, settarismi divisioni territoriali, insomma, per impedire il fallimento di una riforma che sarebbe una sconfitta certamente per il Governo, certamente per la maggioranza, ma ancor più per tutto il Paese. È la nostra grande sfida per l'innovazione istituzionale dell'Italia. È una sfida nel tempo, nel vivo di una crisi economica globale, e nello spazio (nel Nord come nel profondo Mezzogiorno del Paese) perché il marchingegno ideato e anche affinato non si possa trasformare in un grave rischio, in un salto nel buio per il destino economico e sociale dei cittadini, o in un'ulteriore penalizzazione di territori più deboli e già svantaggiati. Il nostro sforzo è per mantenere sempre viva l'unità giuridica, economica e sociale della Nazione e perché tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo della loro residenza, possano godere di pari dignità sociale. Questa è la nostra sfida. Questa è l'essenza e la premessa della nostra democrazia. Signor Presidente, Presidente del Consiglio, ministro Bossi, Ministri, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, oggi in Aula stiamo per realizzare quello che solo fino a pochi anni fa sembrava ai più impossibile: il federalismo fiscale. E lo stiamo facendo in un clima completamente cambiato dal passato. Il tema del federalismo fiscale, da oggetto di aspre critiche e da spettro della lacerazione del Paese, da bestia nera del pensiero politico ed intellettuale di questo Paese, si è oggi trasformato nell'argomento principe del dibattito sulle riforme. È stato accettato anche da chi non lo condivideva e lo contestava. E non se ne parla solo in politica: ne parlano gli studiosi di economia, si scrivono saggi e testi, si organizzano convegni, si susseguono scambi di opinione sui quotidiani, se ne parla sui posti di lavoro e nei luoghi di ritrovo. Tutti parlano di federalismo e tutti hanno qualcosa di positivo da dire in proposito. Chiedono l'approvazione del federalismo le associazioni di categoria, i commercianti, gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori, gran parte dei sindacati. Anche il Capo dello Stato ha definito ineludibile l'approdo al federalismo fiscale. Di questo siamo contenti. Oggi, però, non ci importa rivendicare il fatto che siamo stati noi per primi, della Lega Nord Padania, a parlare di federalismo. Ci interessa, invece, che questo progetto sia condiviso il più largamente possibile. E su questa linea ci siamo mossi anche in fase di discussione di questo provvedimento. Potevamo approvarlo con i soli voti della maggioranza. Abbiamo, invece, da subito cercato il dialogo anche con i colleghi dell'opposizione. Devo dire che grazie all'atteggiamento responsabile di tutti siamo riusciti a discutere questo provvedimento senza tensioni, senza scontri tra maggioranza e opposizione, cosa che invece è sempre avvenuta in passato. Voglio dunque ringraziare tutti i colleghi del Popolo della libertà, del Movimento per l'autonomia, ma anche i colleghi dell'opposizione, del Partito democratico e dell'Italia dei valori. È la prima volta nella storia di questa Repubblica che una riforma così importante per lo Stato non è stata motivo di contrapposizione politica. Anzi, in Commissione, il testo è stato approvato senza nessun voto contrario. Non era mai successo. Abbiamo, invece, lavorato con pazienza e con attenzione per arrivare ad un federalismo condiviso, in grado di essere utile a tutto il Paese. Quel federalismo che da tempo il Nord reclama a voce alta, ma che ora viene richiesto dai cittadini che vivono nelle Regioni meridionali. È da tempo ormai che al Nord la gente non è più disposta a pagare tutte le tasse allo Stato centrale e vedere che molto spesso questi soldi vengono spesi male, se non addirittura sprecati. Anche al Sud, in molti si sono stancati di un assistenzialismo fine a se stesso, sterile, improduttivo, che in tanti anni non ha cambiato le cose. La gente, onorevoli colleghi, non si fida più di chi amministra i suoi soldi, il ricavato delle sue tasse, da lontano, dal buio dei palazzi, nel segreto, dove è più facile imbastire favori, dove si causano sprechi senza che nessuno veda niente, soprattutto senza che ci sia un responsabile. La stragrande maggioranza dei cittadini ci chiede forme di governo più concrete, più vicine al territorio in cui vivono. Ed è per questo motivo - ne sono convinto - che riusciremo non solo ad approvare, ma anche ad attuare il federalismo fiscale, perché il popolo che convintamente lo vuole ce lo chiede ed in politica la volontà popolare vince sempre. Con il federalismo fiscale cambieremo l'impostazione di questo Stato, abbandoneremo per sempre il centralismo e l'assistenzialismo che negli anni, è giusto ricordarlo, hanno fatto sì che il nostro Paese producesse il più alto debito pubblico in Europa, uno dei più alti uno dei più alti nel mondo, un vero record negativo, una zavorra che ha bloccato interi settori produttivi, che ha frenato la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Con il federalismo fiscale le tasse non andranno più tutte allo Stato centrale, non andranno più tutte a Roma, non sarà più Roma a decidere su tutto e non sarà più Roma a decidere per tutti. Andremo finalmente a dare autonomia finanziaria ai nostri Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni. Ciò avverrà senza costi aggiuntivi per i cittadini. La pressione fiscale complessiva dovrà ridursi ad ogni trasferimento trasferimento di funzioni dallo Stato alle autonomie. Diretta conseguenza dell'attuazione del federalismo fiscale sarà dunque la diminuzione del prelievo fiscale: lo Stato chiederà meno tasse. Abbandoneremo per sempre il criterio della spesa storica: lo Stato, fino a oggi, trasferiva di più a certi Comuni e meno ad altri; introdurremo invece il criterio dei costi standard: tutti avranno le stesse risorse e non ci saranno più Comuni o Regioni di serie A o di serie B. Tutto ciò sarà fatto gradualmente, in modo non traumatico, usando anche meccanismi perequativi per permettere a tutti di adeguarsi alle nuove norme. Gli amministratori locali però saranno obbligati a rispettare i vincoli di bilancio. Bloccheremo gli sprechi: i sindaci, i presidenti di Province e di Regioni che sprecheranno denaro pubblico saranno commissariati e non potranno più essere eletti. Non ci saranno per loro prove d'appello: chi sbaglia paga. La finiremo per sempre con opere pubbliche iniziate e mai finite, con le assunzioni per i voti di scambio, con l'abuso di auto blu, con ospedali o strutture sanitarie costruiti e mai utilizzati. Questo non potrà più accadere, sarà solo un triste ricordo del passato. Il risultato di questo lavoro è una riforma destinata a durare negli anni ed a sopravvivere ai Governi, che rilancerà questo Paese sia dal punto di vista politico che amministrativo. Decentrando i poteri dello Stato e responsabilizzando gli amministratori locali riusciremo a garantire servizi migliori ed i benefici si faranno vedere da subito: avremo scuole più curate ed un miglior servizio sanitario, rilanceremo le infrastrutture locali garantendo anche una miglior gestione del trasporto pubblico. un ulteriore vantaggio: saranno i cittadini a valutare l'operato dei propri amministratori; nessuno potrà più dire «la colpa non è nostra» e scaricare responsabilità a qualche anonimo dipartimento ministeriale. Saranno così i cittadini con il loro voto a premiare o bocciare chi ha il compito di gestire i soldi che pagano in tasse. Daremo un'immagine migliore di noi anche al di fuori del nostro Paese. Gli altri Paesi europei ci guarderanno con più rispetto. Nessuno ci potrà più irridere a causa delle nostre inefficienze, come è avvenuto con lo scandalo dei rifiuti di Napoli. Con l'approvazione di questo provvedimento raggiungeremo così gli altri Paesi europei che da tempo si sono strutturati in un sistema federale; ne cito alcuni: la Spagna, la Svizzera, l'Austria, il Belgio, la Germania, la Gran Bretagna. Noi come loro. Onorevoli colleghi, lo avevamo promesso in campagna elettorale: questa sarà la legislatura delle riforme, questa sarà la legislatura del cambiamento. È dunque grande la soddisfazione mia e di tutti i senatori del Gruppo della Lega Nord Padania nell'approvare oggi, a soli pochi mesi da questa nuova esperienza di Governo, il federalismo fiscale, che realizzeremo - lo ricordo a tutti - senza dividere, senza penalizzare nessuno, nell'interesse dell'intero Paese e delle generazioni future.

Signor Presidente, onorevoli senatori, signori rappresentanti del Governo, Presidente del Consiglio, poche volte mi è accaduto nella mia ormai lunga esperienza parlamentare di avvertire così forte la responsabilità di un voto. Certo, incide la qualità straordinaria della questione, nel senso di *extra ordinem*, rispetto al consueto dei lavori parlamentari. Si dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione, sostituendo all'attuale un altro impianto istituzionale, che riguarda sotto il profilo delle prerogative fiscali l'intero sistema delle autonomie (Regioni, Comuni, Province). Abbiamo anche la consapevolezza della parzialità di questa riforma, visto che qui e insieme non discutiamo anche della Carta delle autonomie, cioè del riordino dei poteri, delle funzioni e dunque delle risorse da assegnare alle autonomie. Lo faremo presto, ha assicurato ieri il ministro Calderoli. Noi attendiamo, - voglio sottolinearlo - non sarà un'attesa paziente perché avvertiamo quanto mutilo sia per questo motivo il nostro ragionare di oggi. Mi capita - penso che capiti a tutti - di pensare in chiave di metafora e mi è successo in questi giorni di pensare a questa riforma come a una di quelle bandiere che lo scalatore pianta sulla cima della vetta conquistata. Dopo, quel luogo non è più lo stesso: la presenza dell'uomo lo cambia, ma quella bandiera è esposta a tutti i venti e sorge in un luogo inesplorato e non ha, a sorreggerla, niente intorno. Sta, come direbbe il ministro Tremonti, in una terra incognita: appunto. Ieri il Ministro ha qui riferito circa una nostra pressante richiesta, quella di conoscere l'impatto della riforma in termini economici e finanziari. Preoccupazione legittima l'ha definita il Ministro; più che legittima - direi io oggi - nell'incalzare degli effetti di una crisi che - temiamo - durerà qualche anno, come qualche anno durerà l'emanazione dei decreti legislativi e, quindi, il compiuto inveramento di queste riforme. Il ministro Tremonti ci ha risposto, con chiarezza, che non è possibile oggi rispondere alla domanda che abbiamo posto, perché troppe sono le variabili in gioco, ma che sarà possibile, volta per volta, valutare l'impatto economico di ogni singolo decreto legislativo. La risposta non ci ha soddisfatto - lo sapete - ma soprattutto essa ha riproposto con forza la questione che sin dall'inizio abbiamo sollevato, cioè quella del ruolo del Parlamento nell'attuazione del federalismo fiscale. È la questione sulla quale abbiamo più insistito e rispetto alla quale non abbiamo avuto ancora risposte sufficienti e rassicuranti, perché a valutare e a controllare i decreti legislativi e, a questo punto ministro Tremonti, a valutare l'impatto economico di ciascuno di essi, sarà un organo - la Commissione bicamerale - che non ha un potere in più rispetto alle Commissioni permanenti. Un Parlamento disarmato, dunque, di fronte ai testi del Governo e rispetto all'impatto economico che quei testi porteranno con sé. La nostra preoccupazione è una preoccupazione seria. Ieri il presidente Pisanu ha affermato che prima vengono le scelte e poi vengono i conti, restando il fatto che se i conti non dovessero tornare si ritornerà sulle scelte, e ha ribadito che l'approvazione del provvedimento è un atto di fiducia nel dialogo che si svilupperà in Parlamento: appunto. Ciò richiederebbe che il Parlamento avesse, con la Commissione bicamerale, una sua propria speciale forza nei confronti, non del Governo e non di questo Governo, ma dei Governi che si succederanno in questi anni. Non è così con questo testo e mi auguro che così non sarà ancora, ma che il percorso successivo veda un ripensamento serio, profondo, radicale su questo punto. Un non conosciuto, quindi, e ove non conoscibile non governabile. Quella bandiera, però, è anche investita dal vento impetuoso delle politiche centralistiche del suo Governo, presidente Berlusconi. Non sono però quelle dettate, come pure accade in altri Paesi europei, dalla necessità di fronteggiare la crisi con politiche neocentralistiche. Mi riferisco a ben altro; mi riferisco al taglio dell'ICI che ha privato di risorse essenziali i Comuni per una scelta strumentalmente demagogica, socialmente inutile, dannosissima per le municipalità e cui non corrisponde ancora l'impegno del Governo alla restituzione. *(Applausi dal Gruppo PD).* Mi riferisco anche al decreto-legge che ha sostituito lo Stato alle Regioni su capitoli definitivi come scuola e sanità o ancora, per citare la lettera di ieri dei Presidenti delle Regioni, alla gestione del Fondo sociale europeo; e potrei continuare. Certo è che il federalismo fiscale si colloca in un quadro di compatibilità con le scelte politiche centralistiche, che lo infragilisce e solleva dubbi veri e perplessità sulla sua sorte finale. Una contraddizione politica che la coalizione di maggioranza è in grado di reggere per la sapienza distributiva con cui concede qualcosa a ciascuno degli associati, ma che non può rassicurare il Paese e che mostrerà presto la corda. Eppure, qualcosa di davvero positivo è accaduto in questo *iter* parlamentare. Cose significative per il nostro Gruppo e per il nostro partito, che è innanzitutto una grande forza nazionale, rappresentante e governante in tutte le aree del Paese, al Nord, al Centro, al Sud. Siamo una forza che, insieme alle altre che componevano il centrosinistra, nel 2001 ha voluto la riforma del Titolo V della Costituzione. E - voglio dirlo per stroncare forse definitivamente, me lo auguro, tanta favolistica - era lo stesso testo approvato prima in Commissione bicamerale e poi in Aula, a larghissima maggioranza. Siamo la stessa forza che contribuì a sconfiggere con il *referendum* la successiva riforma del centrodestra e che oggi è stata a pieno titolo nella discussione parlamentare ed ha capovolto la filosofia di quel testo governativo sul federalismo che partiva da un impianto egoisticamente centrato sulle Regioni ricche e fondato sulla suggestiva tentazione che veniva offerta a quelle Regioni di trattenere sul proprio territorio la ricchezza prodotta, tutta la ricchezza prodotta, incurante di ogni ragione del Mezzogiorno e dei suoi cittadini, delle disparità territoriali, dei *gap* infrastrutturali, delle disuguaglianze nell'accesso ai diritti sociali di tanta parte del Paese. Non è più così nel testo che abbiamo discusso in Aula. Ce lo riconoscono gli osservatori ed anche gli studiosi più critici. Ciò che abbiamo con la nostra proposta e con la nostra fatica contribuito grandemente a determinare è un modello potenziale di federalismo, che è in grado di fondare, se lo vorremo, una nuova unità nazionale. Un federalismo ispirato al principio di sussidiarietà, che prevede che verticale sia la perequazione e dunque tutela le aree più deboli, che prescrive uguali diritti e asseconda il processo per ottenerli con una gestione affidabile, trasparente e verificata nei costi, che muove verso la responsabilità degli amministratori, principio tanto più utile nel Mezzogiorno per sconfiggere gli antichi mali e per promuovere e premiare le amministrazioni virtuose. Se lo vorremo, certo. Una forza riformista non può indietreggiare rispetto a questo. Ha il dovere e la responsabilità di collaborare perché questo sia. Ma, soprattutto, ha il dovere di vigilare perché questo sia. Siamo all'inizio di un percorso che sarà lungo e ancora da fare. E sarà il risultato finale a determinare il nostro atteggiamento definitivo; niente, da questo punto di vista, è scontato. Ma nel frattempo siamo stati, per questa ragione e a pieno titolo, con la nostra proposta, nel percorso parlamentare abbiamo sbriciolato - me lo lasci dire, presidente Berlusconi - il *cliché* dell'opposizione riottosa e incapace di proposta, a dimostrazione che, quando c'è la disponibilità del Governo e della maggioranza, noi ci siamo. Io non so se si replicherà, per esempio sulla giustizia. Ma quello che è chiaro, a questo punto, è che la faccenda dipende dal Governo e dalla maggioranza, che dal Governo e dalla maggioranza dipende la possibilità di costruire consenso intorno a riforme che servano al Paese. Ma si è anche rovesciata una prassi oppositiva, in quest'Aula e in quelle Commissioni che hanno lavorato al federalismo fiscale. Non è «no» a tutti costi, sempre, se si è all'opposizione, com'è stato in passato per noi, ma anche, identicamente, per voi nella scorsa legislatura. Questo torna a farci riflettere ancora su un tema che è molto chiaro: se il federalismo fiscale passasse solo con i voti della maggioranza, se avesse solo il segno e la cifra della maggioranza, e forse, ancora di più, la cifra soltanto di una delle forze che compongono la maggioranza, cosa accadrebbe? Qualora cambiasse domani la maggioranza di Governo, si cambierebbe nuovamente il federalismo fiscale e questo Paese, che ha bisogno di crescere, di rafforzarsi, di modernizzarsi, farebbe la fine di una pallina da ping pong che rimbalza inutilmente su un tavolo deserto. Inoltre, è passato sin troppo tempo dal momento in cui abbiamo approvato la riforma costituzionale, di intervenire. Il nostro partito ha molti ringraziamenti da fare a tutti coloro i quali hanno lavorato, a tutti i colleghi del mio Gruppo, ma specialmente lasciatemi ringraziare i componenti delle tre Commissioni che si sono impegnati, il nostro relatore di minoranza Vitali, i componenti del Comitato ristretto, a cominciare dai nostri responsabili nelle tre Commissioni. Abbiamo anche da fare

nelle Commissioni e in Aula, ma anche in mille conversari, in mille incontri. Speriamo di trovarlo ancora più attento nelle prossime occasioni.

Le sue parole ci hanno sorretto e confortato nella scelta, rafforzandoci nella fiducia. che annuncio il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, colleghi, desidero iniziare il

che ha portato avanti un lavoro a 360 gradi consultando tutti gli enti locali, tutte le realtà sul territorio: mi riferisco al ministro Calderoli, al ministro Fitto, al ministro Bossi, che ha partecipato personalmente a molte sedute delle Commissioni, e al ministro Tremonti, che ha fatto la sua parte, così come si conviene a uno che fa il Ministro dell'economia e delle finanze all'altezza della situazione e non l'apprendista stregone che deve dare a tutti i costi i numeri Siamo ad una svolta importante nella storia dell'ammodernamento della nostra Repubblica, perché finalmente riusciamo a conciliare, come due facce della stessa medaglia, il federalismo costituzionale con il tema dell'autonomia delle risorse, cioè il federalismo fiscale. Con senso di responsabilità abbiamo voluto scegliere come punto di partenza una riforma della Costituzione, quella del Titolo V, che non avevamo condiviso e non avevamo votato, perché ci siamo resi conto che se le riforme non camminano appaiando la strada delle leggi dello Stato che attuano le norme della Costituzione, difficilmente si può arrivare a un obiettivo che cambi la realtà di questo Paese. Questo è lo sforzo che abbiamo fatto con grande senso di responsabilità perché non avevamo condiviso inizialmente né la riscrittura dell'articolo 114 della Costituzione né quella dell'articolo 119, di cui questa legge dello Stato è l'attuazione. Entriamo ora in una fase in cui il principio di responsabilità, di razionalizzazione della spesa e di spostamento delle risorse crea il grande cantiere di un federalismo solidale, responsabile, trasparente. Non avremo più amministrazioni in cui si spende a piè di lista perché tanto qualcuno alla fine paga, ma avremo amministratori che dovranno procurarsi le entrate e misurare la loro capacità di amministrare le spese perché

con una battuta, è una sorta di cambiamento del costume che porta ad un «pago, vedo, voto», perché finalmente tra l'amministratore ed il cittadino ci sarà un rapporto che li legherà sulla base di quello che si fa. Si razionalizzerà la spesa, e questo finirà per eliminare le pratiche inefficienti, perché non ci sarà più qualcuno che le paga ma sarà l'amministratore che le porta avanti che dovrà risponderne. È proprio per questo che la parola federalismo è stata una delle più avversate nella storia della nostra Repubblica, dapprima quando si parlava di semplice decentramento e poi quando diventò federalismo; avversata da parte della politica, avversata dalla burocrazia, avversata dai centri di potere romano che pensavano che tutto si potesse fare per la periferia quasi come se si elargissero elemosine o favori al Mezzogiorno e si lusingassero contemporaneamente gli amministratori delle zone più ricche del Paese. È questa la vera svolta: quella che prepara un'amministrazione rinnovata, veloce, moderna, che possa rispondere alle necessità del cittadino e che sarà la prima risposta che daremo alla grande crisi economica che attanaglia il pianeta e di cui risentiamo ovviamente anche noi. Una pubblica amministrazione che risponda alle esigenze del cittadino e delle imprese, che si muova con la velocità con cui dovrà muoversi l'economia per riprendersi è la prima grande risposta che il Governo dà al Paese con questo provvedimento per cercare la strada vero cambiamento. Che ci piaccia o no, credo che lo spostamento delle risorse - lo sa bene il Ministro dell'economia e delle finanze - ridurrà le disponibilità dello Stato e quindi sarà necessaria una cura dimagrante, in un Paese in cui sino a pochi anni fa - non so se esista ancora - viveva un ufficio stralcio per le pensioni di guerra o si ricostituivano i Ministeri bocciati dai *referendum*, cambiando il nome nel giro di poco tempo, perché il potere centrale impediva il cambiamento e lo snellimento dello Stato che invece deve muoversi su livelli equiordinati, quelli previsti dall'articolo 114 della Costituzione, che faranno del nostro un Paese diverso da quello che è ora. La spesa, lo abbiamo garantito nelle norme di chiusura del provvedimento, razionalizzandosi, dovrà fornire gli stessi servizi senza crescere i servizi stessi al fruitore, probabilmente nel tempo potremmo anche avere il beneficio di una spesa minore. L'invarianza della pressione fiscale dovrà essere una cura che, attraverso il mantenimento del Patto di stabilità e di crescita, dovremo mantenere. Si è a lungo dibattuto per sapere a chi giova questo provvedimento: alla Lega - molti hanno scritto così porta a casa una norma pensando di aver fatto una buona cosa per un pezzo del territorio? Non l'abbiamo fatto per questo. Noi riconosciamo al movimento e al partito della Lega Nord di aver avuto un ruolo fondamentale nel porre all'attenzione del Paese, dei Governi e del Parlamento questo tema, ma rivendichiamo anche al partito del Popolo della Libertà di aver stretto un patto con la Lega e con gli italiani e di aver svolto una campagna elettorale nella quale abbiamo preso questo impegno con gli elettori, ed oggi comincia questo cammino. Lo diciamo perché vogliamo un'Italia una e federale, un'Italia che vive delle sue diversità,

la perequazione e la solidarietà non possono essere elemosina che si dà a chi è rimasto indietro, ma contributo concordato per un patto di crescita; allo stesso modo la competitività non può essere la corsa folle di 20 Regioni e di alcune migliaia di Comuni che non hanno le stesse capacità, e rischiano di far deragliare tutto il convoglio se non si capisce che o certe cose si fanno insieme, mettendo tutto il Paese in condizione di arrivarci, o non serviranno all'Italia e la divideranno. Questo è lo spirito con il quale stiamo andando nella direzione che vi dico. Abbiamo cercato di lavorare a tutte le esigenze possibili, come si può fare in una legge delega: non ci sono investimenti. Questa non è una legge che che reca stanziamenti; non c'è da portare a casa un contributo per il proprio territorio. C'è da portare a casa una struttura diversa e più moderna delloStato, delle Regioni, delle Province e delle aree metropolitane. Lo abbiamo fatto pensando ai Comuni, da quelli di montagna a quelli di confine; abbiamo previsto i piani speciali d'intervento e la garanzia dell'esercizio dei diritti fondamentali e dei livelli essenziali. Abbiamo pensato alle isole e ai loro grandi problemi, a cominciare dalla Sardegna e dalla Sicilia,

rivendicando un ruolo della politica non come mezzo di posizionamento tattico, ma come strumento per lo sviluppo del Paese e per la ripresa delle imprese. Concludo questo mio intervento annunziando il voto orgogliosamente favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà, signor Presidente del Consiglio, nel nome della battaglia che ci ha portato a fare, nel nome del successo che lei ha avuto alle elezioni politiche e del processo di cambiamento che con il suo Governo abbiamo cominciato a portare avanti

rappresenta la forza del cambiamento, di quel cambiamento che non ha paura del nuovo, quando il nuovo significa il meglio per il nostro Paese. Nel nome di questa forza, nel nome di questo Presidente del Consiglio e dei consensi ricevuti, dovremo andare avanti su questa strada, per fare sempre più grande il nostro Paese e per essere sempre più vicini agli italiani.

Signor Presidente del Senato, signori responsabili del Governo, signor Presidente del Consiglio,

di un intervento concordato, che rappresenta quattro senatori. Le motivazioni di questa difformità rispetto al nostro Gruppo parlamentare stanno se da un parte appare certamente un'indeterminatezza del quadro generale di questo provvedimento - ma, come dice il ministro Calderoli, tutto è migliorabile - dall'altra, non possiamo non sottolineare come nell'articolo 24 ci sia un rispetto degli Statuti delle Regioni speciali.

Signor Presidente, la storia del movimento repubblicano affonda le sue radici nelle autonomie locali, nel federalismo, ma soprattutto nell'unità del Paese. Quella, però, che ci viene presentata è oggi una delega generica, perciò totale, che demanda l'effettivo potere normativo per una riforma costituzionale così importante e rilevante per il futuro del Paese al Governo, e quindi ai burocrati, che detteranno effettivamente le norme. Il Parlamento, in modo sbrigativo, viene espropriato di una sua propria funzione nel determinare le risorse e le modalità con le quali si finanzia il fondo perequativo e tutto il resto. una riforma centrale per gli aspetti politico-istituzionali del Paese viene avviata in modo superficiale, senza una Carta delle autonomie, senza un approfondito esame di quell'unico organo costituzionale che detiene la sovranità. Ancora una volta, le nostre sorti e le nostre scelte destinate a incidere nella nostra vita per decenni sono affidate alle segrete e manipolate decisioni di una burocrazia irresponsabile. Scelta frettolosa, quindi, e infelice nel merito per noi, perché nella legge delega manca ogni riferimento vero alla solidarietà, che deve essere la premessa irrinunciabile di qualsiasi riforma costituzionale. Altri Paesi europei - un esempio per tutti la Francia - stanno scontando gli esiti negativi di frettolose riforme federali e non abbiamo avuto risposte al federalismo perché, al federalismo per cosa e al federalismo con quali soldi. L'attuazione degli obiettivi enucleati nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione dovrebbe essere compito di tutti: della Repubblica, delle Regioni a Statuto speciale, delle Regioni a Statuto ordinario, dei Comuni e delle Province. Così non è, perché - è solo un esempio, ma quanto importante - le Regioni a Statuto speciale restano lì con tutti i loro problemi e privilegi e nello sforzo solidaristico non sono coinvolte. È per questo che tale progetto non è né unitario né federalistico, è solo un pasticcio, per cui non può votare a favore chi, come i repubblicani, appartiene ad una tradizione politica secolare, che ha sempre sostenuto il più ampio decentramento nel rispetto dell'unità solidaristica della Nazione.

ringraziare tutti voi, ringraziare l'Assemblea per il clima di grande collaborazione che è stato posto in essere da tutti i colleghi sin dal lavoro in Commissione.

Mi auguro che questo clima di confronto radichi sempre in noi la convinzione che la centralità del Parlamento è essenziale perché si possa trovare un momento di sintesi reale politico-parlamentare tra maggioranza e opposizione. Il confronto, il dialogo, la sintesi devono avvenire in Parlamento: questo è il luogo istituzionale voluto dagli italiani; questo è il luogo deputato a fare in modo che il legislatore possa lavorare al meglio nel confronto e nel rispetto di una coalizione nei confronti dell'altra. Questo è un momento importante di questa legislatura, sono felice di poter assistere a questo momento e di poter presiedere questa Assemblea, e di questo vi sono grato. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, desidero richiamare l'attenzione dell'Aula problematiche da cui, in varie Regioni d'Italia, il mondo dell'agricoltura è afflitto a seguito delle gravi avversità atmosferiche e delle copiose piogge

i lavori sono terminati più tardi del previsto e non mi sarei avventurato in un'atmosfera del genere. Mi rendo conto; però, il problema desidero comunque rappresentarlo, perché è urgente e grave. e delle problematiche che in questo momento soffre ulteriormente un comparto già in crisi, come quello dell'agricoltura, a seguito delle gravi avversità atmosferiche e delle copiose piogge degli ultimi giorni. Ne hanno fortemente risentito numerosissime aziende agricole e tante aziende zootecniche. Danni ingenti sono stati prodotti alle colture, in particolare alle coltivazioni orticole, interi raccolti sono andati distrutti. I riflessi del maltempo si sono abbattuti anche sulla viabilità, e in particolare su quella rurale, come pure sui fabbricati rurali, oltre che, come ho già detto, sui terreni agricoli. In Liguria, nel Veneto, in Emilia-Romagna, in Basilicata, in Sicilia, in Campania il comparto agricoltura - notoriamente segnato dalla crisi, i cui esiti non vengono alleviati dalla persistente disattenzione del Governo - è oggi in ginocchio: vi sono vasti territori nel Paese, già drammaticamente colpiti da eventi calamitosi in un passato non lontano, che hanno conosciuto in queste ultime nuove fasi di preoccupante emergenza. Parlo, tra gli altri, dell'Agro-Nocerino-Sarnese, nel Salernitano, con particolare riferimento

a parte, signora Presidente, il Comune di Sarno, che rappresenta un caso a se stante. La tragica alluvione del 1998 produsse morti e distruzioni: in 137 persero la vita, e altri lutti si ebbero a Siano e a Bracigliano, oltre che a Quindici, in Irpinia, e a San Felice a Cancello, nel Casertano. A me pare che rispetto ad una situazione così grave e così diffusa in vasta parte del Paese, in primo luogo con riguardo alla più urgente emergenza del comparto agricoltura, ma poi anche rispetto ai danni registrati alla viabilità e all'abitato, sia indispensabile che il Governo assuma urgenti provvedimenti, valutando la necessità di proclamare - ove necessario - lo stato di emergenza. Sarebbe opportuno che il Ministero delle politiche agricole, per quanto di propria più diretta competenza, promuova accertamenti ai quali conseguano adeguati e risolutivi provvedimenti.

Approfitto della presenza del ministro Bossi per rendergli noto che Muammar Gheddafi, due ore fa, ha chiesto di coinvolgere Osama Bin Laden in un dialogo di pace per cercare in qualche modo di trovare una soluzione politica al terrorismo internazionale. settimana prossima, a partire dalla Commissione affari esteri, sarà in discussione il Trattato di amicizia Italia-Libia. Mi domando se si debbano dare cinque miliardi del contribuente a qualcuno che vuole combattere, o forse no, magari riabilitare anche il terrorismo internazionale altrui, visto e considerato che noi abbiamo già riabilitato quello libico con dei soldi pubblici. Quindi, invito i presenti a prendere in considerazione anche queste ultime dichiarazioni di Gheddafi, ma soprattutto chiedo che, quando si arriverà al dibattito in Aula, ci sia grande pubblicità, pari a quella che è stata data oggi al provvedimento sul federalismo